Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Sottosegretario, continua il percorso riformatore di questa maggioranza e di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare.

Con il provvedimento in esame intendiamo passare da un intervento di legislazione d'emergenza ad un intervento sistematico e strutturale. vorrei ricordare l'estinzione del reato per condotte riparatorie: si tratta di un istituto che, sul piano deflattivo, porterà una serie di reati, il cui perseguimento assorbe tempo, lavoro e mezzi, ad essere risolti nel tiro di poche battute. Questo sarà possibile, ovviamente, per i reati di nessun allarme sociale, perché si tratta di reati a querela della persona offesa, in cui quest'ultima, una volta avuto risarcimento totale, è più che soddisfatta. Inoltre, si interviene sui riti alternativi, strumento assai utile per un sistema giudiziario congestionato come il nostro: tali tipi di soluzione delle controversie devono essere rinforzati perché assicurano giustizia in maniera rapida ed efficace. Relativamente all'impugnazione, la delega contenuta nel disegno di legge in esame attribuisce al Governo la facoltà di intervenire, senza incidere sulle garanzie della difesa, per razionalizzare alcuni meccanismi che avevano portato all'abuso di tale strumento difensivo. Viene stabilito finalmente un termine certo per lo svolgimento delle indagini preliminari e per la decisione di archiviazione o rinvio a giudizio a carico dei magistrati: è il segnale di un cambiamento culturale affinché tutti gli attori che prendono parte al processo rispettino regole e tempi, anche per tutelare i diritti della difesa. Ricordo, ancora, gli aumenti di pena per i reati di furto e rapina. Le modifiche al regime delle intercettazioni sono finalizzate a impedire la diffusione delle intercettazioni che non hanno alcuna rilevanza penale. Inoltre, si puniscono le condotte in cui le intercettazioni vengono carpite fraudolentemente, per offendere la reputazione altrui. Durante il lavoro di Commissione si è giustamente deciso di rimandare ad una più compiuta e ponderata trattazione la riforma della materia delle notificazioni: la finalità acceleratoria delle norme inizialmente immaginate, infatti, non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, mettendo a rischio la conoscibilità, da parte dell'imputato, dei capi d'imputazione contestati. Per quanto riguarda il sistema carcerario e la vita dei detenuti, il disegno di legge mira ad una semplificazione delle procedure: vengono dettate norme per il contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. Per incoraggiare la rieducazione delle persone in carcere si è positivamente deciso di propendere per una revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative. Ispirate al recupero e alla reintegrazione sociale dei detenuti sono anche le misure di incoraggiamento alle attività di giustizia riparativa e di valorizzazione del lavoro e del volontariato. Infine, si è stabilito di procedere con un adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale. Sulla prescrizione, infine, si interviene prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo il primo grado

si coniuga la risposta alle esigenze processuali di termini più lunghi con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Questa riforma è il frutto di una mediazione raggiunta in Commissione giustizia grazie all'approccio collaborativo di tutti i Gruppi parlamentari. Punto essenziale dell'intero provvedimento è la tutela dell'imputato e il rispetto della garanzia costituzionale di un equo processo, che non può in alcun caso configurarsi come un procedimento dalla fine incerta e quanto mai vaga. La ragionevole durata del processo e le garanzie a tutela dell'imputato sono punti cardine di uno Stato di diritto liberale

i quaranta articoli che compongono il complesso provvedimento all'esame del Senato recano importanti modifiche dell'ordinamento penale, dal punto di vista sia sostanziale che processuale. In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, l'Atto Senato 2067 interviene anche sulla cornice sanzionatoria di alcuni reati, come il furto, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso. È su questo che concentrerò il mio intervento, pur consapevole che l'attenzione politica e mediatica è rivolta ad altro, in particolare al gigantesco tema della prescrizione e di come assicurare il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi in un ordinamento come quello italiano che prevede - diversamente da altri - l'obbligatorietà dell'azione penale. Ma altri colleghi sono già intervenuti ed altri ancora lo faranno. Passando specificamente al contenuto sostanziale del Atto Senato 2067, ricordo qui l'articolo 1, che inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, che consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose e pericolose del reato. Si tratta, ovviamente, solo dei reati perseguibili a querela di parte, comunque soggetta a remissione. L'intento è quello di consentire, laddove possibile, la riparazione del danno e, quindi, la dichiarazione dell'estinzione del reato. Ove ciò non sia possibile, trattandosi di un fatto che non dipende più dalla volontà dell'interessato, si dovrà comunque procedere nella medesima maniera. È evidente che l'intento è prevalentemente di tipo deflattivo, per evitare che i reati di piccolo cabotaggio intasino l'attività dei lavori degli uffici della della procura e dei giudicanti, che a qualcosa di più importante debbono dedicarsi. L'ottica, dunque, è quella di migliore l'efficienza del sistema penale italiano, ovvero di concentrare le risorse, in particolare quelle umane, laddove serve. L'articolo 3 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio.

ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sul fronte della condotta incriminata e dilatandola considerevolmente perché è stata ricompresa, come da più parti si chiedeva (ricordo note campagne di incentivazione), anche l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell'erogazione, di altra utilità, oltre che di denaro. Restava il problema della cornice sanzionatoria che nel testo in discussione trova ora una più completa previsione: il disegno di legge al nostro esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Ma quello su cui vorrei attirare l'attenzione sono soprattutto gli articoli da 4 a 6. Con tali articoli infatti si realizza una forte stretta su scippi, furti in casa e rapine: i reati più avvertiti dagli italiani, quelli che minano la sicurezza della propria casa e la possibilità di muoversi liberi in strada. Sono i numeri a dare sostanza alla percezione dei cittadini: la frequenza dei furti, una casa svaligiata ogni due minuti, l'aumento esponenziale con il raddoppio dei furti in dieci anni. I dati Censis ci dicono che erano 110.887 nel 2004, ma già nel 2013 erano saliti a 251.422: ben il 127 per

Cresce, contemporaneamente, anche l'attenzione delle Forze dell'ordine nei confronti di questo reato. Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per furti in abitazione 15.263 persone per cento rispetto al 2004), di cui 1.366 minori, e sono state arrestate 6.628 persone. I detenuti per furto in abitazione e furto con strappo erano 3.530 nel 2014, con una crescita del 131 per cento rispetto al 2007. L'aumento dei reati che turbano la quiete domestica porta a un aumento delle preoccupazioni della gente comune. Era necessario intervenire ed è stato fatto. In questo testo si sono previsti aumenti di pena mirati soprattutto ad evitare che scippatori, ladri e rapinatori, una volta arrestati dalla polizia, magari dopo importanti fatiche investigative, Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, ovvero furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e rapina L'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva dall'attuale anno a tre anni e la pena pecuniaria, nel minimo, dagli attuali 309 a 927 euro e, nel massimo, dagli attuali 1.032 a 1.500 euro. La disposizione inasprisce, inoltre, anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624*-bis* del codice penale. Significa che il minimo edittale sale dagli attuali tre a quattro anni - e tutti sappiamo cosa ciò significhi - con pena massima prevista di dieci anni, se il reato è aggravato dalla violenza sulle cose o dalla destrezza o dalla presenza di più persone ovvero dalla presenza di una sola ma travisata o da una persona che si finge pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando, perciò, della fiducia della vittima. sempre con riferimento all'articolo 624*-bis* (furto in abitazione o con strappo), il disegno di legge n. 2067 aggiunge un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, concorrenti con una o più

alle circostanze aggravanti. L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Nel caso delle circostanze aggravanti elencate dal suddetto articolo, il reato di furto - quello per così dire è punito con la pena della reclusione da due a sei anni, aumentando anche in questo caso il minimo edittale. Infine, l'articolo 6 interviene sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni La disposizione inasprisce, inoltre, anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624*-bis* del codice penale. È una risposta adeguata e sufficiente? Forse per altre forze politiche presenti in quest'Assemblea no; ma fornire ai magistrati strumenti efficaci, garantire procedimenti penali solerti è indispensabile per restituire ai cittadini un maggior senso di sicurezza. È un dovere insopprimibile per lo Stato. E questo disegno di legge è sicuramente un passo utile in tale direzione. signor Ministro, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge vogliamo riformare un capitolo fondamentale per il buon funzionamento della macchina statale, erogatrice di servizi per i cittadini quali la disciplina del processo penale. Una necessità per il nostro Stato di diritto evidenziata con fermezza da più parti, non solo da parte di alcuni soggetti, talvolta anche portatori di interesse personale, ma davvero dalla stragrande maggioranza degli utenti della giustizia. Proprio il settore della giustizia, sotto il profilo dei tempi e delle risposte di certezza e a causa del ridotto finanziamento, da un lato, e di una scarsa progettualità di investimento sugli aspetti più logistici, dall'altro, non riesce a dare risposte e servizi efficienti ai cittadini. Per cui, velocizzare il processo penale era uno dei temi che maggiormente hanno mosso i lavori della Camera, prima, e della 2a Commissione del Senato, successivamente. Certamente durante l'*iter* di formazione di questo disegno di legge ci sono stati momenti di confronto tra sensibilità politiche diverse all'interno del Parlamento: questa è la dimostrazione più evidente della complessità, allorché si introducono aspetti che incidono profondamente sui meccanismi della giustizia, e conseguentemente sulla vita reale di tantissimi cittadini, di arrivare davvero ad una norma che sia chiara, precisa e immediatamente applicabile senza alcuna forma di perplessità nell'interpretazione. ha il compito di trovare un equilibrio politico di sintesi delle varie istanze, rappresentate anche durante le audizioni svolte, cui ha partecipato la maggior parte dei più rappresentativi esponenti della magistratura, dell'avvocatura, della carta stampata e del mondo dei media. Vorrei evidenziare alcuni punti qualificanti del provvedimento oggi al nostro esame, che rappresentano proprio tale equilibrio. Abbiamo previsto un inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio, come i furti e le rapine, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Sono state aumentate anche le pene edittali per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. In tema di intercettazioni, si è cercato giustamente di limitare quelle intercettazioni captate fraudolentemente, e soltanto al fine di ledere l'onore delle persone. Si è inteso, quindi, rafforzare il principio della garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche, in conformità al dettato costituzionale, nella effettuazione e nella gestione del materiale intercettato, specialmente con riguardo alle persone occasionalmente coinvolte dai procedimenti di indagine. Sono state dettate misure per la semplificazione del processo penale, specificamente per razionalizzare le possibilità di proporre appello avverso alle decisioni del giudice e conseguentemente per accorciare i tempi della giustizia. Vorrei ricordare che con questa normativa stiamo dando attuazione a un percorso riformatore in cui abbiamo tenuto conto delle forti indicazioni provenienti da istituzioni e organismi europei. Mi riferisco in particolare alla giustizia riparativa, che mancava come principio culturale nel nostro ordinamento, per la quale è stata conferita una delega al Governo circa l'ampliamento della facoltà di controllo di informazione della persona offesa. Tale aspetto si inserisce in una più ampia delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, in cui si presta attenzione anche al recupero e al reinserimento dei minori detenuti, delle donne in carcere e delle detenute madri. Per concludere, mi sembra che il risultato del testo elaborato dalla 2a Commissione del Senato rappresenti un punto di vero equilibrio. Tutto, evidentemente, è perfettibile, specialmente in materie articolate e di dettaglio come quella penale, ma oggi facciamo più di un passo avanti verso un modello migliore e più efficiente di giustizia penale. Presidente, onorevoli colleghi, i lavori che hanno portato la Commissione a valutare positivamente il provvedimento sono la testimonianza di uno scambio fecondo e continuo non solo tra Esecutivo e Parlamento, ma anche tra Parlamento, addetti ai lavori e le diverse figure professionali. avviene proprio perché ci troviamo di fronte a un tema che inevitabilmente richiede la consapevolezza di dover procedere con il metodo del confronto e con l'esame dell'esperienza concreta, senza la possibilità di avere soluzioni precostituite e infallibili. Proprio per questi motivi, ci troviamo di fronte un provvedimento che ha alle spalle una lunga gestazione, la cui la verifica degli effetti e dell'impatto è assolutamente necessaria. Con questo disegno di legge si interviene su materie molto diverse, che vanno dal rafforzamento delle garanzie difensive alla durata ragionevole dei processi, al tema dell'ordinamento penitenziario, affinché i principi costituzionali dell'effettività della pena, compresa la sua funzione rieducativa, e delle garanzie della difesa siano rispettati fino in fondo. Elencando brevemente i punti salienti del provvedimento, vorrei ricordare l'aumento delle pene per i reati contro il patrimonio; la delega per la riforma delle intercettazioni, che mira ad assicurare un uso garantista nel segno della riservatezza del materiale intercettato; le misure per la semplificazione del processo penale, con specifico riguardo alla materia delle impugnazioni; la riforma dell'ordinamento penitenziario, con particolare attenzione alla giustizia riparatoria. Ebbene, tutte queste materie vengono ricondotte a unità nel testo oggi in esame, credendo che contenga soluzioni ragionevoli e ispirate anche al principio di proporzionalità.

Vorrei anche sottolineare quello che sembra un corretto bilanciamento del rapporto tra Parlamento ed Esecutivo per quanto riguarda le deleghe. Le deleghe previste sono necessarie, perché ci troviamo di fronte a prospettive aperte e non abbiamo la possibilità di poter tradurre il tutto in una regolamentazione analitica e di dettaglio. Esse hanno, in prospettiva, una capacità di verifica ulteriore nel ritorno dei provvedimenti del Governo anche all'esame consultivo del potere legislativo. ci sarà ancora occasione di verificare la coerenza dei provvedimenti che l'Esecutivo riterrà di dover prendere proprio sulla base del disegno di legge oggi in esame. Rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre dei mali cronici che tutti conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Il provvedimento in discussione apre a un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione giustizia. Oggi intendiamo mettere le basi per un profondo lavoro sull'organizzazione, sui mezzi, sulle risorse, su una corretta rielaborazione del modo di essere degli uffici e sul sostegno agli operatori. Il Parlamento avrà poi il compito e la responsabilità di verificare se le misure adottate in via legislativa saranno dell'utilità immaginata e se tutti gli attori coinvolti nella riforma dell'universo penale saranno messi nelle condizioni di operare per garantire una giustizia rapida, equilibrata ed efficace ai nostri concittadini. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il disegno di legge in esame costituisce uno dei diversi interventi attraverso i quali in questa legislatura viene affrontato dal Parlamento il tema della giustizia in un'ottica di riforma. L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia hanno rappresentato - e per molto aspetti continuano a rappresentare - il terreno di un aspro scontro politico che, per molto tempo, ha impedito che fossero avviate le necessarie riforme atte a garantire efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese: tanto più si è discusso e ci si è scontrati negli ultimi anni attorno a questo tema, tanto più si è lasciato che le sue disfunzioni più gravi diventassero mali cronici. La giustizia è divenuta in tal modo per i nostri cittadini e le nostre imprese non la sfera a cui rivolgersi per vedere garantiti diritti o dare tutela ai propri legittimi interessi, non la dimensione dove anche il più debole tra i cittadini possa trovare riparo dai soprusi del più forte, ma il simbolo di un calvario da tenere il più lontano possibile dalla propria vita, e questo nonostante il valore della professionalità e delle competenze che operano all'interno del vasto pianeta giustizia. Di tutto ciò è stato il Paese a fare le spese. Oggi il malfunzionamento del sistema giudiziario rappresenta secondo tutti gli osservatori più avvertiti, e soprattutto secondo chi ci guarda da fuori, uno dei più grandi macigni sulla strada della crescita e non ci consente di sedere a pieno titolo tra i nostri migliori *partner* europei. La complessità della giustizia italiana è tale da non poter essere affrontata con un unico intervento riformatore, con un'unica soluzione, con un intervento ritenuto messianico. Quello che invece abbiamo avviato in questa legislatura come maggioranza di Governo e come parlamentari è stato un percorso per tappe, che ha certamente visto lo scambio continuo e proficuo tra Governo e Parlamento. Non ci siamo trovati a esaminare unicamente atti d'iniziativa governativa. governativa. Importanti atti d'iniziativa parlamentare hanno trovato piena legittimazione nel rapporto con il Governo e con il voto parlamentare.

la cosiddetta e tanto attesa depenalizzazione che, proprio al Senato, in Commissione giustizia ha trovato spazio e legittimazione e finalmente è diventata anche un importante strumento di intervento;

che hanno minato e continuano a minare gravemente l'economia italiana. Quello che ci apprestiamo a esaminare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti, principalmente processuali, ma anche di diritto sostanziale. Ricordo l'approccio culturale e tecnico che abbiamo voluto utilizzare: innanzitutto, si è introdotta una sorta di doppio binario culturale. Nel nostro Paese è possibile tenere insieme la sicurezza con le garanzie? Per molti no. Per anni abbiamo visto un conflitto tra queste due dimensioni: i sostenitori della sicurezza contro i sostenitori delle garanzie; chi prestava attenzione alle garanzie trascurava il tema della sicurezza. In questo disegno di legge, finalmente, si crea un ponte tra la dimensione della sicurezza e quella delle garanzie. E ripeto finalmente: siamo arrivati in ritardo, ma l'innovazione di questo approccio deve essere valorizzata e premiata.

Anche questo doppio binario è entrato tra le norme. E siamo stati molto attenti, meticolosi, nell'evitare che una giusta attenzione al tema delle garanzie potesse minare il tema della sicurezza sotto il profilo, appunto, della lotta alla mafia e al terrorismo. Alcuni esempi molto concreti voglio anticipare in cui il doppio binario (culturale e tecnico-giuridico) ha trovato piena legittimazione: mi riferisco all'articolo 18 del

faccio riferimento, in particolare, a questa disciplina, che è stata molto discussa e alla quale noi riteniamo si debba prestare molta attenzione: «In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di - ben -quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a*), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello». Come vedete, anche qui il principio del doppio binario ha trovato piena legittimazione: c'è una differenza di trattamento per reati comuni e per reati di mafia e di terrorismo. È chiaro che anche il vincolo dei tre mesi per i reati comuni può creare qualche difficoltà. È, quindi, necessario che il Ministero della giustizia - e per questo mi rivolgo al Ministro si organizzi in modo tale, come si sta facendo in questi mesi, da razionalizzare, potenziare e migliorare la capacità organizzativa delle procure, la capacità di dare una risposta in termini di organico e di personale amministrativo,

che dà conto del doppio binario tecnico-giuridico, che è stato - come sapete tutti - pensato e ideato da Falcone e che oggi è una realtà viva all'interno del nostro codice. L'articolo 36 del nostro disegno di legge reca «Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario». Anche questa è una riforma molto attesa; una delega importante che offriamo al Governo, su cui il Parlamento vigilerà ed è tenuto a dare dei pareri. Seguiremo con molta attenzione questo punto di portata innovativa, atteso da tanti e tanti anni e richiestoci dalla società civile, dagli operatori del mondo del volontariato e dell'associazionismo e dagli osservatori europei e internazionali sul pianeta carcere. Ricordo a tutti i nostri colleghi che noi, fino a qualche mese fa, avevamo il problema del sovraffollamento, il male principale che attanagliava il pianeta carcere. Io debbo qui ringraziare il Ministro e il Governo, ma debbo dire anche che un contributo importante l'ha offerto il Parlamento, in particolare proprio il Senato, per fare in modo che il nostro Paese non fosse più attanagliato da questo problema. E la riforma adesso è arrivata. Non abbiamo più il tema del sovraffollamento. La riforma trova spazio e lo trova secondo il criterio del doppio binario. Innanzitutto, proprio al primo comma dell'articolo 36 si presenta bene il doppio binario e si dichiara in modo chiaro, netto e preciso: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,» - il famoso 41-*bis*, sottolineo io di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

le importanti, sottolineo, misure alternative - «sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo» - ecco qui il doppio binario «che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare» - aggiungo a scanso di equivoci - «per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale». Doppio binario c'era e doppio binario rimane; questo punto non viene scansato.

Recita il punto *e)*: «eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari» - ecco qui la garanzia del doppio binario - «in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato». In sostanza, si vuole fare un salto di qualità, che già la senatrice Ginetti nel suo intervento ha ben spiegato. Non si tratta qui di massificare l'intervento. Non si tratta di pensare che tutti i tipi di detenuti siano messi nella stessa condizione. Bisogna puntare a un trattamento sempre più individualizzato e differenziato, che deve però tener conto del tipo di reato commesso. Noi sappiamo che, per i reati di mafia e terrorismo, la caratteristica aggregativa, anche all'interno del carcere, è la filiazione;

i benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, ovvero una categoria molto delicata e importante, che sono i vari *boss* di primo piano, i cosiddetti capi delle varie organizzazioni mafiose. si dice che occorre intervenire, salvo però i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati e, comunque, nei casi di condanna per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

non si è fatta una scelta volta a limitare l'utilizzo delle intercettazioni. Questo punto non è stato ritenuto meritevole di cambiamento da parte del legislatore. Quindi, nessuno può pensare che nel nostro Paese, attanagliato da problemi gravi, come la corruzione e i reati di mafia e terrorismo,

delle intercettazioni, per evitare che una pubblicazione impropria potesse ledere il diritto alla *privacy* dei cittadini. Quindi, la delega che proponiamo al Governo si muove all'interno di un solco ben preciso

Anche su questo sistema, molto invasivo, si è svolta una discussione all'interno della Commissione giustizia e si è utilizzato il principio del doppio binario, seguendo le indicazioni emerse recentemente in giurisprudenza.

che evita che questo strumento realmente invasivo - lo sottolineo - possa sfuggire a un controllo democratico, diventando lesivo della tutela della *privacy* e delle relazioni umane anche di soggetti esterni a quelli indicati come oggetto dell'indagine, e possa diventare strumento improprio di ricatto, anche da parte di un sistema di potere, che nel nostro Paese è spesso sfuggito ai controlli democratici. E, quindi, si è scelto anche qui di seguire un doppio binario.

che la domanda di sicurezza nel nostro Paese possa diventare solo oggetto di convegni o studi, dove ci si straccia le vesti, si dichiara tutti che è necessario intervenire e dove spesso si fa a gara a chi ritiene che bisogna essere molto vigorosi

tenendo in piedi quella proporzionalità che la nostra Costituzione ci chiede quando si deve intervenire in tema di pene. E i relatori hanno presentato un emendamento che va in questa direzione,

un limite che riguardava la durata della pena. Ebbene, si è deciso - e il Senato ha apprezzato la volontà della Camera - di aumentare la reclusione da sei a dodici anni.

perché tale uso è stato sempre possibile sin dal 1992 quando il 416-*ter* è entrato all'interno del nostro sistema. Così era, così rimane e così sarà: l'uso delle intercettazioni è legittimo e l'aumento della pena non ha spostato il suo utilizzo, non rileva intorno a tale utilizzo che permane e resta importante, perché nel momento sorgivo della democrazia non devono esserci interferenze di tipo mafioso. La libertà del voto deve essere assolutamente garantita e, quindi, il legislatore fa bene a fare una scelta rigorosa per impedire che ci possa essere, appunto, un'interferenza da parte delle organizzazioni mafiose.

oggetto di innovazioni, spostandosi sul piano accusatorio, ma mantenendo alcuni residui del modello inquisitorio, per cui la durata ragionevole del processo non è riuscita più a trovare piena cittadinanza. C'è stata una rivisitazione di tutte le fasi processuali e si è riusciti a trovare quelle soluzioni che sono in grado, anche qui, di tenere in piedi quel doppio binario culturale di cui parlavo prima: più garanzie e allo stesso tempo più sicurezza per i cittadini ad avere processi veloci, ben fatti e ben strutturati. Occorre evitare lo sconcio

l'autorevolezza e la forza di una democrazia, incapace di decidere velocemente e stabilire se una persona è realmente innocente o colpevole. Quindi, cari colleghi,

ma deve essere riconosciuto che il Parlamento, in sintonia con il Governo, sta compiendo una cosa degna di un Paese che finalmente ha il coraggio di affrontare l'argomento, ossia riformare il sistema giustizia e fare dei passi avanti realmente innovativi.

si debba riconoscere una cosa: il Movimento 5 Stelle aveva ragione. Quando ha fatto la battaglia sull'articolo e ha detto in tutti i modi in quest'Assemblea e alla Camera che era una norma sbagliata, aveva ragione.

Ci sono voluti due anni per riconoscerlo e i danni compiuti non sono riparabili, perché l'abbassamento della pena - il regalo che è stato fatto a chi si accorda con la mafia per avere i voti - rimane malgrado l'aumento che oggi

E questo, pervicacemente, non lo si è voluto affrontare e, quindi, cosa si fa? Si usa lo specchietto per le allodole: dopo aver regalato lo sconto di pena a tutti quelli che ne usufruiranno - e saranno tanti - adesso

una vergogna, una macchia che resterà negli anni a venire su questo Governo e la sua maggioranza. A questo non si è posto rimedio nemmeno con questa norma.

Signor Ministro, cose così importanti che attengono alla libertà dei cittadini vanno discusse in questa sede davanti a tutti, assumendosi prendendosi la responsabilità delle scelte che si fanno.

mette a rischio. È vero che lo salva per i condannati all'ergastolo per mafia, ma apre la porta a possibili interpretazioni che non vorremmo vedere, perché non vogliamo assistere a un regime carcerario differente per i condannati per mafia. Non vogliamo veder fare questo regalo alle mafie.

punto 3, e immaginate come sono scritte queste norme. Stiamo parlando del più potente strumento di indagine in questo momento a disposizione delle procure, che può essere attivato soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Ebbene, esclusi i reati di mafia e terrorismo, per attivare le indagini in via informatica ci vuole la flagranza di reato, ovverosia non potrà mai essere attivata, perché non vi sarà la certezza della flagranza del reato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. puntavate e che si voleva ottenere: legare le mani alle procure. Ma non basta: abbiamo riempito le procure di atti burocratici e chiusure entro tre mesi delle indagini dopo la scadenza dei termini, che è un

un testo degli studi universitari - il famoso saggio di Santi Romano - che parlava dei destinatari delle norme giuridiche. Chi sono i destinatari di queste norme? Per chi sono scritte queste norme? Sono scritte per i cittadini di questo Paese?

percorsi a ostacoli su percorsi a ostacoli. Ci chiedono norme efficaci e voi cosa fate? Legate le mani alle procure, togliendo loro uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla corruzione. Se poi il sospetto è di

che, attraverso le indagini della magistratura, si ricatta qualcuno? Se qua c'è qualcuno che ricatta altri, si tratta dei corrotti che hanno accesso alle strutture marce dello Stato, ad apparati che fanno indagini e a intercettazioni senza avere l'autorizzazione della magistratura, che servono non a portare a processo,

è uno scandalo questa norma! E non venite a dire che serve per combattere la delinquenza diffusa, che è stata invece favorita dai vostri atti. Dopo ben tre decreti svuotacarceri vi siete accorti che in questo Paese l'arroganza dei delinquenti, anche quelli comuni, anche i più spiccioli, anche di quelli di strada, è arrivata alle stelle.

E il giorno prima nel centro della Sicilia, a Barrafranca, hanno sparato colpi di fucile contro la casa di un altro carabiniere. Qui la criminalità rialza la testa perché sa che può godere di ampi margini di impunità, i margini che voi avete garantito con i vostri svuotacarceri, che hanno liberato 28.000 condannati; 28.000 condannati, che stanno facendo banchetto a dispetto dei poveri cittadini del nostro Paese, delle persone perbene. impuniti! E voi ora cosa fate? Alzate le pene per cercare di rimettere in galera quei 28.000 che avete liberato?

Si vuole agire per impedire quelle indagini che portano dritti al cuore della corruzione del nostro Paese, ma senza danneggiare le indagini contro la mafia. Ebbene, sappiate che importanti studiosi del fenomeno dicono da anni che non c'è mafia senza corruzione; che ci può essere corruzione senza la mafia, ma non c'è la mafia senza corruzione. E voi cosa fate? Indebolite la lotta alla corruzione quando questa è il primo problema di questo Paese. Qui non esiste alcun problema di *privacy*.

Ma la nostra *privacy*, quella dei deputati e dei senatori dell'opposizione, è messa a rischio dalle indagini illegali e non da quelle della procura, perché noi dalle procure non abbiamo nulla da temere. Abbiamo da temere dai vostri apparati, quelli foraggiati dalla Ebbene, noi voteremo contro questo provvedimento. Voteremo contro perché è un provvedimento ignobile, che non dà giustizia a questo Paese e che favorirà ancora una volta la corruzione e la mafia che su questa pasce.

anche attraverso un confronto serrato, cercando di rappresentare le diverse sensibilità su temi controversi, oggetto di molti ed articolati interventi con giudizi diversi e a volte opposti. Gli interventi più critici si sono concentrati sul tema della prescrizione argomentando obiezioni forti rispetto alle scelte operate. Non voglio eludere la questione, ma credo occorra ribadire e sottolineare la complessità delle norme in esame che toccano molteplici aspetti. Il provvedimento cerca di migliorare l'apparato normativo a disposizione per perseguire con maggiore efficacia alcuni reati, modificando e affinando strumenti, disciplinando le fattispecie oggetto di intervento, tenendo insieme le ragioni delle vittime dei reati e la tutela di chi è imputato. Il provvedimento è corposo e tocca molti aspetti rispetto ai quali colmiamo anche un vuoto normativo. È una risposta utile e dà il senso di un processo riformatore che va avanti e che dà il segno di una determinazione a proseguire anche rispetto alla delega sulla riforma complessiva del processo penale. Vorrei soffermarmi e ripercorrere alcune norme significative di questo provvedimento. Come ho detto

al contenuto del provvedimento, voglio citare in particolare alcune norme come l'articolo 1, che inserisce il nuovo articolo 162-*ter* del codice penale, che riguarda i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, che favorisce la riparazione del danno e la dichiarazione di estinzione del reato. C'è un evidente intento deflattivo, onde evitare che i reati di piccolo cabotaggio intasino l'attività degli uffici della procura e dei giudicanti. Si tratta di una direzione auspicata da tempo, su cui finalmente si va ad operare concretamente, perché è evidente che c'è tutta una serie di reati che ingolfano l'attività degli uffici giudiziari e contribuiscono a creare delle inefficienze della giustizia che producono danni enormi su questioni di maggiore interesse e di maggiore attenzione che dovrebbero avere, con un processo giusto e in tempi rapidi, risposte molto diverse dalle attuali. L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendo il quadro sanzionatorio. Già nel corso della legislatura è intervenuta una modifica che ha ampliato la gamma delle condotte ricadenti nella previsione della norma e ridotto la pena. Con questa ulteriore modifica vi è un inasprimento della sanzione con la pena della reclusione da sei a dodici anni rispetto a quella prevista attualmente da quattro a dieci L'articolo 4 interviene sui delitti di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo della pena detentiva da un anno a tre anni, oltre ad elevare la pena pecuniaria. La nuova disciplina interviene sul quadro sanzionatorio delle condotte aggravate, come pure sulle circostanze attenuanti concorrenti con quelle aggravanti del furto di cui all'articolo 625, che non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, evitando che possa essere vanificata la credibilità della pena per queste fattispecie.

è poi un blocco di norme che interviene sulla prescrizione (gli articoli dal 7 all'11) e che hanno costituito il cuore di tanti interventi critici in quest'Aula. Un intervento di carattere normativo

e per il reato di violenza sessuale e di *stalking* se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza. In questo caso la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Con tale disposizione si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia all'inizio di questa legislatura. Si dà pertanto una risposta a un tema che è purtroppo di grandissima attualità.

cronache. L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Si interviene con norme che fissano termini certi in tema di richiesta di autorizzazione a procedere e di deferimento della questione ad altro giudizio; in caso di ragioni di impedimento delle parti, un'ulteriore ipotesi è la richiesta di rogatorie all'estero. Oltre a norme sempre in tema di prescrizione, vorrei citare l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale in tema di regime di procedibilità di alcuni reati e per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici e riabilitativi. Anche in questo caso, credo si colga nel segno intervenendo su una materia molto sensibile, oggetto di discussione, di confronto e di attenzione su un tema molto delicato. C'è poi anche l'importante articolo 13, che contiene la delega per la disciplina del casellario giudiziale. Molto importante, poi, è la delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Da sottolineare, ancora, il tema delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: si dovrà garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. dunque - che pure ho ripercorso in maniera sintetica - che cerca di cogliere le esigenze di innovazione e di evoluzione della sensibilità del Paese e che persegue obiettivi molteplici, come colpire con maggiore efficacia alcuni reati, tutelare maggiormente le vittime di taluni delitti, migliorare l'efficienza dell'apparato normativo che disciplina il processo penale. Sul tema controverso della prescrizione vi sono due esigenze contrapposte, entrambe meritevoli di tutela: evitare che le inefficienze della giustizia consentano di vanificare il perseguimento di reati attraverso la prescrizione; dall'altra, evitare che le stesse inefficienze siano causa di una penalizzazione del cittadino, presunto innocente fino a sentenza definitiva, sottoposto ad un processo interminabile, senza ottenere una sentenza che possa accertare la sua innocenza o la sua colpevolezza. È vero: si può sempre rinunciare alla prescrizione, ma, con i tempi dilatati dei processi che arrivano a situazioni abnormi, paradossali,

Le norme che introduciamo in materia si muovono dentro questo solco segnato dalle opposte esigenze indicate, entrambe - lo ripetiamo - meritevoli di essere garantite. Tuttavia, la riforma del processo penale in delega al Governo potrà consentire una migliore tutela per il diritto del cittadino ad un processo giusto, che consenta di esplicare appieno il proprio diritto di difesa, in tempi certi, senza che la prescrizione assuma, nel bene e nel male, un ruolo così influente come quello di oggi. finché la prescrizione sarà al centro del dibattito e sarà un istituto utilizzato per cercare di far valere l'una o l'altra delle esigenze citate, credo che saremo sempre nella condizione di una difficoltà grave e non saremo in grado di garantire un processo giusto.

insopportabile per il cittadino la lunghezza di questa fase. Mi riferisco sostanzialmente al fallimento della funzione dell'udienza preliminare, che doveva rappresentare un elemento di garanzia del

alla chiusura della fase d'inchiesta, con una ipotesi di reato contestata al cittadino, prima di arrivare davanti all'udienza preliminare può passare un tempo enorme, interminabile. Nel momento in cui si fissa l'udienza preliminare,

In tutto questo enorme lasso di tempo, già dal momento dell'avviso delle indagini, quando viene data l'informazione alla pubblica opinione, si hanno tutta una serie di passaggi: la chiusura delle indagini, la proposta di una ipotesi di contestazione di reato, l'arrivo davanti all'udienza preliminare e il rinvio a giudizio; abbiamo quindi già avuto più sentenze anticipate di condanna. Quella che poi è l'effettiva sede del processo, in cui le parti, di fronte ad un organo terzo giudicante, possono fare valere le proprie ragioni, costituisce oggi una reale garanzia per il cittadino perché, perché, grazie a Dio, attraverso la magistratura giudicante che esercita con professionalità, competenza ed equilibrio la propria funzione, il cittadino stesso ha la possibilità di far valere le proprie ragioni. solo al primo grado di giudizio, però, trascorre un lasso di tempo incredibile. Pensare di colmare l'ingiustizia che si produce in questa lunghissima fase attraverso il ricorso all'istituto della prescrizione significherebbe aggiungere

penale. Proseguiamo oggi con questo passaggio nel processo riformatore e modernizzatore della giustizia. Naturalmente tutto questo non dovrà essere disgiunto da un deciso cambio di rotta in termini di risorse a disposizione del sistema, altrimenti le riforme rischiano di rimanere sulla carta. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà. l'opinione pubblica e la società, sulla necessità di mettere mano ad una riforma della giustizia, di aggiornarla e di adeguarla. Tutti sappiamo quanto sia difficile, soprattutto quando ci si trova sono presenti sensibilità diverse, mettere d'accordo le parti politiche e trovare un punto di coesione che inevitabilmente è sempre al rialzo. Con il provvedimento che stiamo discutendo oggi

rappresenta una delle sfide più impegnative per questo Governo, per questa maggioranza e per il Paese intero. Sappiamo bene come una serie di malfunzionamenti che riguardano proprio la macchina della giustizia siano profondamente connessi con una serie di malfunzionamenti del sistema Paese e del sistema Italia, che non riguardano soltanto il tema della maggiore tutela dei diritti dei cittadini ma lo stesso funzionamento del nostro sistema sociale. Riguardano la capacità dell'Italia di essere attrattiva rispetto, ad esempio, agli investimenti internazionali; di essere un Paese che funzioni superando quell'ampia serie di mali che, dalla corruzione alla più generale mancanza di regole, alla incapacità di vedere nel sistema giudiziario un effettivo luogo di tutela dei diritti della persona, mette in crisi o rappresenta un limite importante rispetto al fatto che l'Italia sia un Paese considerato affidabile secondo criteri nuovi, moderni, aggiornati, esigenti, e quindi uno Stato di diritto in piena regola. Il disegno di legge che stiamo esaminando è corposo e complesso perché tale è la materia oggetto di esame e profonda è l'opera di riforma che si vuole approvare. Ci sarebbe da discutere per mesi, data l'estensione e l'importanza delle modifiche che si vogliono apportare all'ordinamento penale, ma vorrei ripercorrere brevemente i punti imprescindibili del provvedimento. Nei 40 articoli troviamo norme relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie, la riforma della prescrizione, l'inasprimento delle sanzioni per reati gravi e odiosi come lo scambio elettorale politico-mafioso, il furto e la rapina; inoltre vengono dettate norme di semplificazione del processo penale e vengono assegnate deleghe al Governo per il riordino della delicatissima materia delle intercettazioni e per l'altrettanto fondamentale riforma dell'ordinamento penitenziario, ispirando le modifiche al tema della giustizia riparatoria. Infine, non viene trascurato neppure il capitolo della semplificazione delle procedure in materia penale, cui è dedicato il Titolo II del disegno di legge. Si è poi presa la decisione di sospendere di un anno e sei mesi il decorso della prescrizione dopo il primo grado altrettanto dopo l'appello. A questo proposito, grazie al lavoro della Commissione, in Senato si è adottata una modifica importante del testo che ci è arrivato dalla Camera, riducendo da due anni a

si soddisfa l'esigenza processuale di disporre di termini più lunghi per il giudizio e nel contempo si mantiene la natura garantista dell'istituto. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto di stampo liberale, equilibrato, come previsto dal codice del 1930, seppur con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini (aggiornamenti dovuti rispetto al proliferare di questi reati nella nostra epoca, che è diversa rispetto a quella in cui sono state concepite queste norme) per le fasi d'impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Sul fronte del procedimento penale vorrei ricordare particolarmente la disposizione che impone termini certi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con il coinvolgimento del procuratore generale presso la corte d'appello. Quest'ultimo dovrà anche vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, con eventuale illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse. Per quanto riguarda la delega sulle intercettazioni, vorrei sottolineare il rilievo attribuito al principio della garanzia della riservatezza delle comunicazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, in conformità con l'articolo 15 della Costituzione; un articolo che, in verità, negli ultimi tempi è stato regolarmente violato, con le difficoltà conseguenti a trovare i responsabili di tali violazioni perché non si faceva un'operazione preventiva sulla verifica

a tutta una serie di episodi che sono assolutamente collaterali e poco c'entrano con gli atti processuali, che riguardano più la la vita privata degli indagati o che si riducono, a volte, a fenomeni mediatici di *gossip*. Questo sicuramente non rende un favore alla giustizia e ai contenuti del processo stesso. Da questo punto di vista, sembra assolutamente positiva l'attenzione alla tutela delle intercettazioni a carico delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, anche rispetto alle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Sarà punito, finalmente, anche chi diffonderà intercettazioni illegali per danneggiare la reputazione altrui. Infine, la Commissione ha avuto il merito di dettare criteri direttivi precisi e puntuali relativi alle intercettazioni con i captatori informatici, il cosiddetto virus *trojan*, che è stato utilizzato fino a questo momento dagli investigatori senza regole precise, mettendo chiaramente in discussione e a dura prova anche il diritto alla *privacy* di ogni cittadino. Di primario rilievo appaiono anche alcuni profili della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Mi riferisco all'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, di cui si intende facilitare l'utilizzabilità.

all'individuazione di attività di giustizia riparativa e all'incremento e alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e di volontariato per i detenuti, tutti intesi come momenti qualificanti per il percorso di recupero sociale degli stessi. Molto positivo è anche il rilievo attribuito alle esigenze educative dei detenuti minorenni e agli specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri. Il lavoro in Commissione è stato intenso e non si può negare che vi siano stati momenti di vivo confronto tra le varie anime politiche della maggioranza e delle opposizioni. La discussione, però, ha sempre rappresentato l'occasione per raggiungere un punto d'intesa più alto rispetto alle posizioni di partenza, trovando soluzioni condivise, che non intaccavano l'efficacia delle misure immaginate. Credo, quindi, signor Presidente, che questa esposizione abbia dato contezza della complessità di questo provvedimento, ma anche della volontà di riformare delle parti del nostro ordinamento che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene e, soprattutto, in tempi ragionevoli. A questo proposito, signora sottosegretaria Chiavaroli, questo non ci esime dal dover necessariamente provvedere a dare le dotazioni strutturali agli uffici giudiziari, perché si possano portare avanti più velocemente e in maniera più efficace i processi. A parte i problemi della prescrizione, che sono problemi di altra natura, quando la giustizia in un Paese civile funziona e riesce a dare delle sentenze in tempi brevi, questa è anche una spia dell'efficienza stessa del sistema. Ma questo non si può fare se non diamo alle procure, ai tribunali e agli uffici giudiziari le strutture e gli uomini adeguati per poter funzionare. quindi la volontà precisa di andare a riformare queste parti del nostro ordinamento, che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire, attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene, ma anche una reale possibilità di recupero e di riabilitazione attraverso il sistema carcerario. L'insieme di tutti i provvedimenti raccolti all'interno del disegno di legge che stiamo discutendo oggi in Assemblea credo rappresenti un fatto veramente significativo. Poi sicuramente la discussione in Assemblea metterà a fuoco alcuni elementi che meritano un ulteriore approfondimento e probabilmente portano con sé la necessità di svolgere riflessioni ulteriori, insieme al Governo. Credo tuttavia che la completezza di questo provvedimento rappresenti un punto di riferimento all'interno di questa legislatura e che, anche per il futuro del nostro Paese, questa riforma contribuirà a dare competitività al Paese e certezze ai cittadini, indipendentemente dal ruolo che ricoprono nel momento in cui sono sottoposti ad un procedimento giudiziario.

il disegno di legge che stiamo discutendo oggi in quest'Aula - se la maggioranza consentirà che la fisiologica discussione su un testo alquanto complesso avvenga è senza ombra di dubbio un provvedimento assai articolato, che tocca molti dei punti nevralgici della giustizia penale: si va dalle modifiche al codice penale a quelle al codice di procedura penale, sino ad arrivare alle riforme dell'ordinamento penitenziario, incidendo su materie quali la prescrizione dei reati (tema che è stato per mesi all'ordine del giorno su tutti i *media*), ovvero (altro tema caldo) la delega per la riforma delle intercettazioni. Si sarebbe indotti a pensare che si sia finalmente posto rimedio all'endemica condizione di inefficienza, quasi di decozione, del sistema della giustizia penale. Ma così non è; basti pensare alla famigerata riforma dell'istituto della prescrizione. I faticosi lavori svoltisi in Commissione ci hanno consegnato un testo per alcuni aspetti incostituzionale, ma soprattutto lesivo del fondamentale diritto dei cittadini ad ottenere giustizia; un testo sul quale non posso esimermi dall'esprimere gravi perplessità. Molti sono gli aspetti di criticità che si possono evidenziare e che forniscono la cifra di superficialità ed approssimazione dell'intervento normativo che la maggioranza vuole spacciare come la svolta risolutiva. Vorrei tuttavia soffermarmi soltanto su alcuni aspetti che ritengo di particolare rilevanza, non solo giuridica, ma per le ricadute in termini di effettiva tutela dei diritti dei cittadino. Penso, ad esempio, all'emendamento dei relatori che ha reintrodotto la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. che tale sentenza segna il limite massimo di operatività dell'istituto: in altre parole, dopo la sentenza di primo grado il processo penale può, in astratto, durare all'infinito. Questa previsione, oltre a violare il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, non tiene in alcuna considerazione un dato fondamentale e univoco delle statistiche giudiziarie, in base al quale è la fase delle indagini preliminari quella in cui matura circa il 70 per cento delle prescrizioni. Di questo, però, la maggioranza non ha tenuto alcun conto. Tra l'altro, la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, per quello che mi pare d'intendere, mal si concilia con le disposizioni successive, che ne prevedono la sospensione al deposito della motivazione della sentenza di primo grado e, quindi, al deposito di quella di appello. In buona sostanza: se la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado, che senso ha prevederne la sospensione nelle fasi successive? Così concepito, l'istituto della prescrizione viola altresì il fondamentale principio della presunzione di innocenza e il diritto della collettività a conoscere, entro il più breve tempo possibile, se un imputato sia colpevole o innocente. Continuo a ritenere essenziale, al contrario, che i processi si concludano innanzitutto in tempi brevi e comunque con una sentenza, che sia di assoluzione o di condanna, che riconosca l'innocenza di colui che sia stato ingiustamente accusato, ovvero la colpevolezza di chi sia stato ritenuto responsabile. Non c'è bisogno che sottolinei che per ciascun cittadino la pena più grave è connaturata alle conseguenze personali, familiari, sociali ed economiche conseguenti alla pendenza di interminabili processi penali. Un siffatto sistema frustra non solo i diritti delle persone sottoposte a procedimento penale nella qualità di indagato o imputato, ma anche quelli delle parti offese, peraltro grandi assenti nelle considerazioni della maggioranza, che si autopromuove riformatrice. parte offesa, come un convitato di pietra, subisce le conseguenze negative di un intervento legislativo farraginoso e contraddittorio. Siamo alle solite, insomma. Il malaffare dilaga, sale nell'opinione pubblica la sete di giustizia e il legislatore che fa? Abdica alla sua funzione, risponde di pancia, giusto ad offrire pannicelli caldi al popolo bue

Ormai non rispondiamo più alle esigenze di giustizia, ma agli *spot* pubblicitari e diamo spettacolo con risse verbali interminabili, che ossessivamente dividono garantisti da forcaioli. Da queste risse il legislatore dovrebbe essere estraneo, altero nella sua funzione e invece ci si cala e ci si imbeve. Il risultato sono questi provvedimenti tampone, che spesso si sommano, di anno in anno, sulla stessa materia e finiscono per mortificare risultato e funzione. Lo dico alla maggioranza e mi appello alla sensibilità giuridica del presidente della Commissione giustizia, senatore D'Ascola: non sono e non possono essere questi né il metodo né la strada. Meglio fermarsi. L'ho già detto in quest'Aula: smettiamo di legiferare, sarebbe molto meglio. Proviamo a vedere, cioè, se cinquecento anni di storia giuridica possono rendere ancora attuale quel Guicciardini del «manco male le sentenze de' turchi», che venivano date a caso e, per il fatto che erano date al buio, accadeva che almeno la metà di esse potesse essere giusta. Un altro aspetto che mi preme evidenziare è quello relativo alla famigerata norma che dispone il raddoppio dei termini di prescrizione per un'*élite* di reati: i reati di corruzione e i reati satellite, considerati gli aumenti di pena introdotti dalla legge n. 124 del 30 maggio 2015, diventano di fatto imprescrittibili. La motivazione addotta a sostegno di tale raddoppio viene indicata nella particolare complessità degli accertamenti necessari alle indagini. Tale complessità, con buona pace del principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, non viene riconosciuta ad altri reati, parimenti gravi e di difficile accertamento, comunque compiuti in danno della pubblica amministrazione. Voglio fare un altro esempio di come la maggioranza si sia ben adoperata per far fronte a problematiche gravi, che incidono pesantemente sulle sorti della vita dei cittadini, di fatto proponendo soluzioni discriminatorie, prive di significato, offensive di un sano buon senso, prima ancora che del pur fondamentale principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che ho più volte invocato. E mi riferisco alla scelta di inserire la prescrizione processuale, in luogo di quella sostanziale, per il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, che gode, in tal modo, di un regime incomprensibilmente differenziato rispetto alle altre ipotesi di omicidio colposo, per le quali continua a valere la prescrizione sostanziale. Uguale trattamento hanno subito alcuni reati ambientali, anche per i quali è stata introdotta la prescrizione processuale. In particolare, mi riferisco ai reati di «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», di «disastro ambientale» e «delitti colposi contro l'ambiente». se è evidente che la *ratio* dell'introduzione di tale disposizione nasce dalla volontà di tutelare situazioni in cui l'evento - di danno o di pericolo - si verifichi a distanza dalla consumazione della fattispecie di reato, è altrettanto vero che, così come proposta, la norma si pone ancora una volta in contrasto con il principio di ragionevolezza a causa dell'arbitraria esclusione di altre fattispecie analoghe a quelle di cui ho detto in precedenza. Superficialità, disattenzione; potrei proseguire ancora a lungo nell'elenco delle distrazioni della maggioranza, ma i tempi mi impongono di limitare questo mio intervento a quanto sin qui esposto, nella speranza che la maggioranza, in un reale dibattito democratico, scevro da preconcetti e logiche di appartenenza, tenga conto delle proposte emendative che, a nome del mio Gruppo, ho presentato. Tra le tante, mi preme evidenziare quegli emendamenti volti a mettere un freno all'illimitata durata delle indagini, attuata tramite il sistema delle proroghe ed il carattere dilatorio del termine di chiusura delle indagini preliminari. La proposta dei Conservatori e Riformisti interviene proprio sulla questa fase, la più critica del procedimento penale, fase in cui i diritti costituzionalmente protetti del cittadino subiscono la più grave compressione. Lo abbiamo fatto tramite l'introduzione del carattere della perentorietà del termine di conclusione delle indagini e la conseguente sanzione dell'archiviazione di ufficio da parte del gip o su istanza della parte ogni qualvolta la procura agisca fuori dai termini perentori così imposti. Questo ritengo sia avere rispetto dei diritti dei cittadini, questo ritengo sia il rispetto del principio e sul rispetto dei principi - permettetemi - non ci possono essere né deroghe né cedimenti. onorevoli colleghi, vorrei brevemente ripercorrere le vicende che hanno portato alla formazione del disegno di legge oggi in discussione. La Commissione giustizia del Senato ha avviato l'esame del provvedimento sulla prescrizione, già approvato dalla Camera il 24 marzo 2015 secondo modalità diverse da quelle individuate dal Consiglio dei ministri, nelle sedute del 9 aprile e del 15 aprile 2015. Nella seduta del 3 giugno 2015 è stato adottato come testo base l'Atto Senato 1844 e la discussione sugli emendamenti si è svolta il successivo 23 giugno. Il 28 aprile di quest'anno la Commissione ha quindi deliberato di procedere alla discussione congiunta anche della riforma del codice penale e del codice di procedura penale per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, già approvata dalla Camera il 23 settembre 2015 (Atto Senato 2067 e abbinati), per il quale sono state svolte anche alcune audizioni, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni. Nella seduta del 4 maggio 2016 è stato adottato un nuovo testo unificato, che riproduce i contenuti degli Atti Senato 2067 e 1844. Dopo un'intensa fase emendativa in Commissione giustizia, il provvedimento risulta composto da 40 articoli e contiene una serie di importanti novità con riferimento particolare a tre profili. Relativamente al codice penale, faccio riferimento all'estinzione del reato per condotte riparatorie e all'innalzamento delle pene per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Rispetto al codice di procedura penale, vorrei sottolineare le norme relative all'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, alla disciplina più rigorosa per lo svolgimento delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, e alla semplificazione delle impugnazioni. Per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento penitenziario sono da accogliere positivamente le norme che incoraggiano l'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno al carcere e le attività di volontariato. Nel dettaglio, vorrei evidenziare solo pochi punti come il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'articolo 3 interviene nuovamente sulla legge n. 62 del 2014, che aveva ampliato la gamma dei fatti punibili (includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione di denaro o di altra utilità). Ora viene inasprito il quadro sanzionatorio, sanzionando il reato di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da sei a dodici anni (anziché da quattro a Il provvedimento interviene anche sulla disciplina della prescrizione: dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, fino ad un massimo di un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza definitiva, sempre fino ad un massimo di un anno e sei mesi. Tale intervento unisce, da una parte, le giuste risposte per garantire la celebrazione dei processi, dall'altra, le garanzie affinché un cittadino non rimanga ostaggio di un sistema giudiziario inefficiente e perverso per anni e anni. Il provvedimento contiene anche una dettagliata delega al Governo per la revisione della materia delle intercettazioni. Tra i principi vorrei solamente ricordare le disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione; l'introduzione di una nuova fattispecie penale per la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente, captate con la finalità di recare danno alla reputazione; una specifica disciplina restrittiva per le per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante i cosiddetti *trojan* (cioè captatori informatici). Per concludere, ritengo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento corposo, necessariamente complesso vista l'ampiezza e la delicatezza delle materie trattate in chiave riformatrice, ma al contempo equilibrato e che possa apportare dei benefici rapidi e concreti al nostro sistema della giustizia e, conseguentemente, a tutti i nostri concittadini e al Paese. dalle agenzie apprendiamo di un presunto ritiro di emendamenti tra quelli già presentati al disegno di legge n. 2067. Siamo nell'impossibilità formale di verificare questa circostanza; al fine di garantire il mio diritto e quello di qualsiasi altro componente di questa

ovvero, qualora prima della fase dell'illustrazione degli stessi, ci si dovesse trovare con la sorpresa di considerare alcuni emendamenti già ritirati senza avere la possibilità di farli propri o aggiungere la firma,

ci siamo trovati a discutere di queste modalità di ritiro di emendamenti, fatto in maniera legittima, ma in una fase non trasparente perché si rischia di non permettere agli altri senatori di avere cognizione dell'intero quadro emendativo. È chiaro infatti che anche le decisioni di voto su altri emendamenti non ritirati possono dipendere dall'effettivo quadro complessivo degli emendamenti. Ci tenevo, quindi, che rimanesse traccia a verbale di questa richiesta da

comunque preannunciato, cosa accadrà, dal momento che non abbiamo notizie ufficiali. La Presidenza lavora sulla base di quanto accade, quando accade, secondo le sue procedure. Gli annunci di stampa ovviamente fanno parte del dibattito. È iscritto È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

si tratta di riforme costituzionali, ci siamo sempre prestati e abbiamo sempre cercato di contribuire a fare in modo che si legiferasse in questo senso.

quella che è la prima parte della Costituzione, che noi riteniamo, in questo momento, non modificabile.

e confusa solo da una parte di questa maggioranza. È un po' come se un chirurgo che opera un tumore o una malattia

tenteremo con ogni mezzo di dimostrare agli italiani che le leggi vanno fatte nel rispetto degli articoli della Costituzione e che bisogna accelerare i processi.

Si continua semplicemente a cavalcare un giustizialismo sospinto da un populismo antisistema a tutti i costi, un giustizialismo che specialmente in quest'Aula e nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è a più riprese manifestato, ultimamente

velocizzare i procedimenti giudiziari e a snellire le procedure in un'ottica di efficientamento del sistema e degli addetti al settore, si gettano le basi

Signor Presidente, colleghi senatori, ci troviamo in questi giorni ad esaminare quello che, a mio avviso, può essere considerato uno dei provvedimenti cardini di questa legislatura, che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. È dunque evidente la portata e l'estrema rilevanza di una norma frutto di un complesso lavoro della Commissione che, dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, ha riesaminato il testo apportando notevoli integrazioni. In questa circostanza, vorrei in particolare soffermarmi su una di queste imprescindibili integrazioni: la regolamentazione dell'utilizzo dei captatori informatici. I captatori altro non sono che *software* occulti che, una volta istallati sui dispositivi tecnologici (*tablet, smartphone, personal computer*) di un inconsapevole utente, consentono di eseguire una pluralità di azioni e di acquisire diversi dati, destinati alla raccolta di prove nelle indagini. Questo strumento investigativo, in uso già da diverso tempo dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, è imprescindibile per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, che ormai basano la gestione e la realizzazione delle proprie attività criminali sull'utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate. Disciplinare, per la prima volta, l'utilizzo di tale tecnologia ha, pertanto, un duplice scopo: da una parte, garantire un sempre più efficace ed efficiente utilizzo di questa strumentazione a distanza nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; dall'altra, far sì che ciò avvenga nel rispetto delle garanzie costituzionali, con una regolamentazione che ne definisca puntualmente i criteri di ammissibilità e le modalità di utilizzo. Difatti, come già ricordato in precedenza dal relatore Casson - che colgo l'occasione per ringraziare dell'attenzione che ha dedicato a questo specifico argomento - la natura di queste tecnologie è tale che, se non opportunamente regolamentate, non lascerebbero traccia delle operazioni effettuate, alterando così la genuinità probatoria dei relativi risultati e rischiando di violare i limiti dell'autorizzazione del È bene, inoltre, ricordare che l'utilizzo dei captatori, consentendo una serie estremamente diversificata di operazioni, come perquisizioni informatiche, geolocalizzazione, intercettazioni ambientali, ambientali, telefoniche e telematiche, acquisizione di dati di traffico, ciascuna potenzialmente oggetto di una specifica disciplina, va a toccare molteplici ambiti giuridici tra loro interconnessi. Il fatto che sia già intervenuta una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione dimostra come le indagini e i processi penali basati sull'utilizzo dei captatori, in assenza di un riferimento normativo specifico, avessero condotto a conflitti insanabili rendendo necessario l'intervento delle sezioni unite. Emerge, quindi, l'importanza dell'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 35, contenente la delega finalizzata a disciplinare l'effettuazione di operazioni intercettative mediante captatore informatico. Tale articolo nel fissare condizioni, termini e garanzie a tutela delle esigenze investigative, statuisce una serie di criteri atti a salvaguardare il diritto di difesa e del contraddittorio sulla prova e, quindi, nel complesso, i diritti dell'imputato e della difesa. Tuttavia, con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, ritengo imprescindibile cogliere l'opportunità del passaggio in Assemblea al fine di rendere più robusta la portata garantista delle disposizioni contenute nella delega. Mi riferisco in particolare alla necessità di rafforzare le misure che che eliminano totalmente la possibilità di delegare la materiale esecuzione di tali operazioni a società private produttrici dei *software* spia, chiarendo incontrovertibilmente che l'utilizzo dei captatori è consentito unicamente sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e con la vigilanza della polizia giudiziaria, nello stringente rispetto dei limiti stabiliti dal decreto autorizzativo del giudice. Sarebbe inoltre opportuno specificare che il trasferimento delle registrazioni possa essere effettuato unicamente verso il *server* della procura o altri *server* posti sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, garantendo che al termine della registrazione il captatore sia disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria. L'articolo in commento, pur nella sua puntualità, non prende in considerazione determinati aspetti che, a mio parere, potrebbero risultare decisivi per garantire un utilizzo tanto efficace quanto equo dei captatori, ossia l'istituzione di un registro nazionale dei captatori e la contestuale individuazione di un processo di omologazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica. Misure che consoliderebbero l'imparzialità e la segretezza delle procedure, assicurando, ad esempio, che siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti per legge, così da garantire che sia l'installazione sia la disattivazione del captatore non alterino i dati informatici e gli elementi di prova memorizzati sui dispositivi in cui è inserito, e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte dal decreto L'attuale formulazione dell'articolo, inoltre, non prevede che, al termine delle indagini, sia riconosciuto alla difesa il diritto di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione, nonché la possibilità di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Infine, sono del parere che la delega debba prevedere la possibilità di elaborare, in fase di attuazione, una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, e per i delitti tentati o consumati da associazioni a delinquere, con specifico riferimento ai delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 416*-bis* e 630 del codice penale, in considerazione della loro particolare gravità. Concludo ribadendo la speranza che il passaggio in Aula possa contribuire a migliorare ulteriormente l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dai relatori, apportando modifiche come quelle che ho esposto finora, così da garantire effettivamente i diritti di tutte le parti coinvolte senza per questo ledere o limitare eccessivamente le possibilità d'intervento delle Forze dell'ordine e della magistratura.

nella seduta di *question time* di domani alle ore 16, il ministro dello sviluppo economico, dottor Carlo Calenda, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: interventi per favorire gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano;

Esiste quindi un turismo terapeutico di cittadini italiani che vanno a curarsi in Egitto in quanto il farmaco è il medesimo, la scatola è la stessa e il principio attivo è lo stesso.

società produttrice lo ha dato ad una società farmaceutica che produce farmaci generici. Io credo, signor Presidente, che il Ministro non conosca questa realtà: il costo per guarire tutti gli affetti da epatite C sarebbe di 60 miliardi

a chiedere al Ministro di venire a rispondere alle tre interrogazioni che ho presentato in quest'ultimo mese sull'AIFA. con quest'intervento continuo oggi in Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. è stato ritrovato, nello scantinato di un immobile della famiglia, il corpo di Giulia Ballestri, di quarant'anni, uccisa a bastonate; per l'omicidio è stato fermato il marito, un noto dermatologo di Ravenna, contro il quale pendono gravi indizi di colpevolezza. Questo fatto conferma che i femminicidi non si consumano solo in una determinata classe sociale, ma sono fenomeni culturali che rispecchiano una concezione di possesso e di potere dell'uomo nei confronti della donna. Giulia è la quattrodicesima donna che abbiamo ricordato fino ad ora in questa staffetta iniziata solo il 30 giugno. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna, che il 47,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*; la gravità delle violenza sessuali e fisiche è aumentata; che sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere; ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica tra uomini e donne, quindi la si può prevenire intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati gli strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Proponiamo nuovamente e con convinzione il nostro appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgo altresì un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.